Comunico che in data 21 ottobre è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della difesa e dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia:* «Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili»

Indubbiamente la richiesta può essere accolta. Ci uniamo naturalmente al cordoglio delle popolazioni colpite e, quindi,

bene.

Signor Presidente, vorrei cominciare facendo dei ringraziamenti non solo al Governo - e in particolare al sottosegretario Bini che ha seguito il provvedimento e alla Presidente della Commissione - ma anche a tutti colleghi. fatto inusuale, ma ritengo sia importante per inquadrare il provvedimento in esame, se si considera che, su un unico emendamento dei quasi 300 presentati, si è vissuto un momento di tensione e divisione, a riprova che su un testo come quello che ci avviamo a convertire in legge c'era comunque una comunione di intenti e di visione da parte di tutti i Gruppi di maggioranza ed opposizione. E non è per maniera che sottolineo come il Parlamento abbia effettivamente migliorato un testo già buono e condiviso da tutte le forze di maggioranza, dando degli spunti in più su un tema che

C'era da intervenire, e il Governo l'ha fatto tenendo presente, ovviamente, un passaggio particolare, che è quello delle competenze delle Regioni. Era quindi necessario un provvedimento quadro che permettesse di

che, disciplinando un nuovo strumento di programmazione statale ai fini del coordinamento relativo alla previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, vuole andare in questa direzione.

il Mezzogiorno, la questione territoriale, la transizione ecologica, le politiche agricole, alimentari e forestali, gli affari regionali e le autonomie. Già il numero dei Ministeri coinvolti dà la misura della complessità necessaria a intervenire, stendere prima stendere prima e attuare poi un piano di siffatta portata. Alla realizzazione del Piano si provvede nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Apro ora una parentesi.

Come approvato dalla Commissione, il Dipartimento della protezione civile provvede in particolare, con cadenza triennale, alla ricognizione e valutazione di un insieme di profili quali le tecnologie anche satellitari volte all'integrazione dei sistemi previsionali, di sorveglianza, monitoraggio e rilevamento nell'ambito, nonché alle esigenze di potenziamento delle flotte aeree, dei mezzi terrestri, delle attrezzature, delle strumentazioni, dei dispositivi di protezione individuale ai fini del rafforzamento della capacità di concorso di concorso statale all'attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, tenendo conto anche di una possibile strategia comune a livello europeo. La Commissione ha introdotto, per far fronte alla capacità di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, il potenziamento dei mezzi terrestri del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Regioni e del volontariato organizzato di Protezione civile qualificato per tale attività, prevedendo inoltre la formazione del personale addetto alla lotta attiva contro gli incendi boschivi, comprese le attività di messa in salvo degli animali coinvolti e all'informazione e partecipazione delle comunità, con particolare attenzione ai territori caratterizzati da un elevato rischio di incendi boschivi. Vorrei sottolineare che anche su questo c'è stata una comunione di intenti fin dalla fase delle audizioni, tant'è vero che il coinvolgimento ha riguardato dalle associazioni ambientalisti fino alla cabina di regia delle associazioni venatorie, ovvero tutti i soggetti, comprese le università e le Forze dell'ordine e le istituzioni, che hanno contribuito molto spesso alla stesura stessa degli emendamenti approvati in Commissione. Al comma 3 si estende anche al Ministero dell'università e della ricerca l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, come previsto dal medesimo comma. Anche in questo caso abbiamo avuto la presenza di valenti esponenti di livello nazionale e internazionale che hanno supportato la Commissione nella fase Il comma 3 aggiunge la previsione che il Ministero per gli affari regionali e le autonomie convochi entro il 30 aprile di ciascun anno la Conferenza unificata sullo stato di aggiornamento dei piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi La Commissione ha previsto che, nell'ambito delle risorse stanziate, il Piano nazionale possa destinare parte dei finanziamenti anche per incentivare sistemi premiali proporzionali ai risultati conseguiti da soggetti pubblici e privati nelle aree in cui sia stata accertata una diminuzione significativa delle aree percorse dal fuoco. Riteniamo questo particolarmente significativo. Il comma 4 dispone per la fase di prima applicazione, previa intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8, l'adozione di un primo Piano nazionale speditivo approntato sulla base della ricognizione condotta dal Dipartimento. La Commissione con un emendamento ha previsto la possibilità di garantire la sicurezza e l'incolumità dei territori dal rischio idrogeologico di strade, ponti e viadotti, nonché di messa in sicurezza e di efficientamento energetico. Il provvedimento infatti, oltre a una parte prevalente relativa al rischio incendi, dedica comunque anche una parte agli interventi di protezione civile. Si inserisce inoltre, come approvata dalla Commissione, la previsione secondo cui, per incrementare l'operatività e la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, per il il numero vacante di posti, è ridotta in via eccezionale a cinque settimane. Anche qui vorrei ricordare che tutti i Gruppi hanno presentato degli emendamenti, a riprova del fatto che su questo c'era un'unità di intenti, così come c'è stata sull'approvazione della norma relativa alla possibilità di un concorso pubblico per 250 posti 250 posti di vigili del fuoco, che possa dare di fatto corpo a quanto previsto dal provvedimento. Sempre su questo, cercando di non abusare della pazienza della Presidente e dei colleghi, è stato istituito con un emendamento un sistema aereo di vigilanza antincendio che possa permettere appunto l'integrazione di questa modalità nella segnalazione degli incendi. All'articolo 2 vengono stanziati 40 milioni di euro per l'acquisto di mezzi operativi e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi,

All'articolo 3 si introducono misure finalizzate a garantire il tempestivo aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco. Vorrei ricordare che, al di là delle singole appartenenze e sensibilità, su uno di questi due articoli, in particolare sull'articolo 3, è stato presentato un emendamento dai relatori, per il quale aspettiamo una riformulazione, che contiamo possa essere accolta in Aula, che va nella direzione che tutti immaginiamo di poter perimetrare e procedere con i divieti

Mi avvio a concludere con un ultimo passaggio relativo all'articolo 3, prima passare la parola al collega. Sono previsti ovviamente aggiornamenti che siano contestualmente pubblicati in un'apposita sezione dei siti istituzionali dei terreni relativi, perché la data del 1° aprile per tutti era eccessiva e serviva una comunicazione più tempestiva. Siamo riusciti a trovare una sintesi e a vederla approvata in Commissione, che speriamo venga migliorata in Assemblea. Il termine di applicazione dei relativi divieti ovviamente rimane lo stesso, mentre è la decorrenza che cambia. Si introduce da ultimo in Commissione la possibilità che le Regioni possano disporre, con propria legge, misure di attuazione di azioni sostitutive in caso di inerzia dei Comuni circa la pubblicazione dell'elenco definitivo dei soprassuoli percorsi dal fuoco; se il Comune non lo pubblica e non lo approva, ovviamente c'è un problema ed è giusto che le Regioni

gli adempimenti di cui all'articolo 10, comma 2, della legge quadro. Gli esiti del monitoraggio sono comunicati alle Regioni ai fini della tempestiva attività dei suddetti poteri sostitutivi. Lascio la parola al collega Quarto per illustrare

oggi in discussione e in approvazione, pur essendo monotematico, è piuttosto complesso. Esso riguarda un problema che ha afflitto l'intera Nazione questa estate, e in particolare le Regioni meridionali, con oltre con oltre 150.000 ettari di bosco incendiati. Anch'io mi unisco al correlatore nei ringraziamenti per l'ottima intesa che siamo riusciti a mettere in campo. Ringrazio l'intera Commissione e gli uffici che ci hanno supportato molto bene. L'articolo 4 reca misure finalizzate al rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi, mediante misure di potenziamento dei piani regionali, nonché stanziando fondi specifici nell'ambito della strategia nazionale per le aree interne, per il finanziamento di interventi volti a prevenire gli incendi boschivi in quelle aree in cui il rischio di incendio è elevato e nei Comuni localizzati nelle isole minori. Sappiamo essere questo un problema estremamente critico per l'abbandono che avviene nelle aree interne. la Commissione ha disposto che, nei piani operativi nazionali attuativi dei fondi strutturali 2021-2027, finalizzati alla sicurezza e all'incolumità dei territori, si tenga conto anche della tutela degli animali. Questo è un altro punto estremamente importante. importante. L'articolo 5 reca misure per il rafforzamento della lotta attiva e dei dispositivi sanzionatori e modifiche alla legge quadro 21 novembre 2000, In particolare, nel comma 1 la Commissione ha introdotto la nuova definizione di incendio di interfaccia urbano-rurale, con cui si intende quella tipologia

Si stabilisce poi che il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi individui, tra l'altro, le aree trattate con la tecnica del fuoco prescritto. Si precisa

devono tener conto delle specificità delle aree protette e di *habitat* di interesse conservazionistico. Si tratta di un altro punto estremamente importante per la tutela dell'ambiente e delle aree protette. Inoltre, nella lotta attiva contro gli incendi boschivi si introduce l'uso delle attrezzature manuali e la tecnica del controfuoco. Quindi, oltre al fuoco prescritto abbiamo il controfuoco. Sono poi rafforzati

della perimetrazione dei soprassuoli percorsi dal fuoco, con gravi problemi che si ripercuotono per divieti in realtà attivati dopo alcuni anni rispetto al fuoco che ha interessato l'area.

previsto dall'articolo 423-*bis* del codice penale, introducendo una circostanza aggravante, quando i fatti sono commessi da coloro che svolgono compiti di prevenzione incendi,

La disposizione prevede inoltre, in caso di condanna, l'applicabilità delle pene accessorie del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, dell'estinzione dell'eventuale rapporto di lavoro pubblico e dell'interdizione all'assunzione degli incarichi legati alla prevenzione incendi, oltre alla confisca obbligatoria, anche per equivalente, dei profitti del reato. L'articolo 7 reca misure ulteriori urgenti in materia di Protezione civile. I commi 1 e 2 recano la ridefinizione delle modalità di svolgimento delle attività istituzionali

Al comma 3 la Commissione ha precisato la proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 ottobre 2023 del termine di durata dei contratti a tempo determinato e delle altre forme di lavoro flessibile, così come previsto dai contratti. Infine, in materia di interventi antropici per la ricostruzione delle superfici boscate, le Regioni possono individuare nell'ambito dello stesso bacino superfici nude, ovvero terreni saldi da sottoporre a rimboschimento compensativo delle superfici bruciate: si tratta di un altro provvedimento estremamente importante. A tal fine, le Regioni possono avvalersi del contributo scientifico di università e ricerca. L'articolo 8 reca disposizioni finanziarie: per la precisione, destina 150 milioni dalla Missione 2, componente 4, del PNRR alle misure di lotta contro gli incendi boschivi, e in particolare per la realizzazione di un sistema avanzato integrato

In relazione al comma 1, nel limite di 150 milioni di euro per la realizzazione della misura di lotta agli incendi boschivi di cui al presente decreto, il Ministero della transizione ecologica valuta, di comune accordo con le altre amministrazioni interessate, di destinare ulteriori fondi del PNRR in favore delle azioni di contrasto alle emergenze incendi, compresi gli interventi di ripristino territoriale, assumendo secondo quanto approvato dalla Commissione - quale ambito di priorità dell'intervento le aree protette nazionali e regionali e i siti Natura 2000 parliamo sempre di una maggiore tutela ambientale - nonché le aree classificate a rischio idrogeologico nella pianificazione di bacino vigente. La Commissione ha precisato altresì che le disposizioni di cui al presente decreto sono applicabili nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Infine, l'articolo 9 dispone che il decreto-legge in esame entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Signor Presidente, membri del Governo, colleghi senatori, il provvedimento in discussione sicuramente entra a far parte di tutti quegli atti necessari per consentire una migliore gestione delle pratiche per la tutela ambientale. E introduce alcuni elementi importanti per il contrasto alla lotta degli incendi: penso - ad esempio - all'introduzione di maggiori risorse per l'acquisto di mezzi necessari per lo spegnimento degli incendi;

come elemento coordinatore nella legislazione fra le competenze Stato-Regioni. Osservando più attentamente il provvedimento, però, vogliamo segnalare come a nostro avviso si rischi di non facilitare, ma anzi di complicare per alcuni versi, la stesura del Piano. Penso - ad esempio - alla composizione del tavolo tecnico elevata presenza di rappresentanti dei vari Ministeri, che rischia una non facile mediazione tra tutte le posizioni. Occorre quindi velocizzare le capacità di azione del comitato tecnico, da una parte pensando a una riduzione della stessa composizione, ma dall'altra coinvolgendo le associazioni agricole (perlomeno quelle più rappresentative a livello nazionale. Nel contempo occorre fare attenzione ad assicurare un efficace coordinamento tra il Piano nazionale antincendio e i piani - ad esempio - di gestione forestale o delle filiere forestali regionali.

La vera prevenzione, colleghi, si fa ribaltando un paradigma fino a oggi introdotto - lo dico con chiarezza - da un'ideologia ambientalista che vuole una gestione della natura completamente autogestita dalla stessa; quella stessa ideologia che si è formata nei salotti buoni di quella *lobby* ambientalista - dico *lobby* con precisione - che ama passeggiare sui sentieri, ma poco o niente sa cosa significa vivere e lavorare in montagna o nei boschi, e per la quale niente si deve fare perché vuole lasciare tutto semplicemente alla gestione della natura. Non è così, colleghi: dobbiamo riflettere su questo aspetto. La prevenzione si fa soprattutto permettendo l'intervento dell'uomo, come hanno fatto per secoli i nostri avi, chi ci ha preceduto. La gestione del bosco deve partire dal suo uso consapevole e sostenibile. ad esempio - qualcosa che potrà sembrare banale: il bosco va tagliato e pulito, non può essere lasciato a se stesso. I vincoli regionali e comunali spesso impediscono una corretta gestione del bosco, senza pensare a tutti i vincoli della soprintendenza che spesso blocca tutto a prescindere. Tutto questo sta provocando un abbandono sempre più importante da parte delle aziende che praticano la selvicoltura. I nostri boscaioli sono sempre più strangolati da una burocrazia asfissiante che non permette loro di svolgere un lavoro già di per sé duro. Occorre quindi rendere il loro lavoro più semplice, per permettere loro di sopravvivere. Il loro lavoro fa prevenzione: non scordiamoci che il loro lavoro è prevenzione. Così come prevenzione viene fatta dalle imprese agricole di coltivazione e di allevamento. Se non permettiamo a tali aziende di sopravvivere - e sottolineo sopravvivere

incendi. Ritornando allora al ragionamento e al paradigma da invertire, significa proprio permettere ai nostri boscaioli, agricoltori e allevatori di svolgere il loro lavoro non solo in quanto tale, ma proprio come primi guardiani ambientali del territorio, soprattutto in territori difficili come quelli montani

Vorrei però fare un'ulteriore riflessione, aggiungendo come ci sia un atteggiamento sbagliato sulla gestione della fauna selvatica, che si basa anch'esso su una visione integralista dell'ambiente. Non è possibile imporre il divieto di caccia nei Comuni limitrofi ai territori dove si è sviluppato l'incendio in maniera netta e incondizionata, come si voleva fare nel dispositivo di legge. Se da una parte possiamo anche capire il divieto nelle zone coinvolte nell'incendio, non si capisce perché si debba interrompere la gestione della fauna selvatica in altri territori, andando di fatto ad aumentarne la presenza spesso nociva per l'agricoltura e per l'ambiente stesso.

all'inizio del mio intervento - elementi sicuramente positivi (le risorse, l'inasprimento delle pene e un maggiore coordinamento), manca comunque una visione della gestione complessiva ambientale, che tenga presente l'apporto positivo

Al di là degli *slogan*, manca una pianificazione vera e integrata della gestione dell'ambiente e dell'uomo che - ricordo a tutti noi - fa parte anch'essa del sistema ambientale. Molto probabilmente, anche questa volta, abbiamo perso un'occasione. *(Applausi)*.

esponenti di Governo, colleghi senatori. la problematica legata agli incendi boschivi è questione di cui il Parlamento già in passato si è occupato.

che il Parlamento, anni fa, decise di affrontare per cercare di dare un'organizzazione normativa regolamentata più logica e più utile soprattutto nella lotta contro gli incendi boschivi

con un approccio sanzionatorio - anche severo - nei confronti di chi aveva dolosamente provocato negli anni passati - ci siamo dovuti rendere conto che anche quella legge, approvata nel 2000, quindi ventun anni fa, purtroppo, non era idonea ad affrontare nel modo corretto una problematica divenuta veramente grave per gli equilibri ambientali del nostro Paese e soprattutto per il nostro patrimonio forestale, che,

una serie di provvedimenti contenuti nel decreto-legge n. 120, varato dal Governo nel settembre scorso,

Si è cercato di porre particolare rimedio ad aspetti già contenuti nella legge precedente, che evidentemente necessitavano di un ulteriore approfondimento, di un ulteriore intervento normativo. alla questione della previsione: come è possibile prevedere che vengano appiccati o comunque che si sviluppino incendi nei nostri boschi? Il tema della previsione è fondamentale. poi la prevenzione: come è possibile prevenire lo sviluppo di incendi? Su questo ho da dire qualcosa; mi pare che anche il collega di Fratelli d'Italia abbia fatto riferimento a questo aspetto, sul quale penso si debba dire qualcosa. Mi riferisco in particolare alla cura di certe foreste e di taluni boschi che, ovviamente, se abbandonati a se stessi, se non curati, possono essere più

Questi tre aspetti sono sicuramente fondamentali per venire incontro ad una esigenza, che non è solo ambientale. Si badi bene che negli incendi muoiono persone e animali

ma bisogna riconoscere che c'è stato un incremento degli incendi e, in particolare, in certi momenti, ad esempio della scorsa estate, c'è stata una diffusione degli incendi spaventosa. Ricordo soltanto i giorni a cavallo Il 31 luglio e il 1° agosto ho percorso l'autostrada A14 "Adriatica", dalla Puglia verso la mia Regione, l'Abruzzo,

non è soltanto un patrimonio forestale e ambientale, è anche un patrimonio culturale e storico per la città. Questo va detto. Certi boschi non sono soltanto un'espressione ambientale da preservare, ma sono anche qualcosa di più,

gli incendi hanno provocato un danno apparentemente irreversibile, anche se si prevedono trenta, quaranta, cinquant'anni per ripristinare il patrimonio boschivo che c'era un tempo, noi dobbiamo applicarci subito e fare in modo che le procedure, le lungaggini, i problemi che la burocrazia talvolta pone siano assolutamente evitati e che i contributi economici per restituire

In quest'Aula spesso si è discusso sulla sussistenza dei requisiti che sono presupposto fondamentale per i decreti-legge. Si è disquisito sulla mancanza degli stessi, sulla

i critici, i requisiti per adottarlo. In sostanza, la scelta della strada della decretazione d'urgenza è sempre stata molto discussa, a ruoli invertiti, a seconda del ruolo che si ha nel Governo. periodicamente, ogni volta che ci troviamo a convertire un decreto-legge, la discussione quasi sempre verte sull'inopportunità della scelta o sulla mancanza dei requisiti. La brevissima discussione che c'è stata fino adesso - che, però, ha visto comunque pronunciarsi anche un rappresentante dell'opposizione - per la prima volta nella mia esperienza di parlamentare non ha eccepito la mancanza del requisito della necessità e dell'urgenza; questo, a mio avviso, perché tutti abbiamo chiaro in mente quanto è successo questa estate: il dramma vissuto in tutta la nostra Penisola, i danni enormi, la sofferenza di animali e persone. nel dubbio che qualcuno ancora non sia convinto dell'opportunità di questa scelta, voglio ricordare alcuni titoli di giornale: «Incendi e desertificazione. Andati in fumo 150.000 ettari di bosco». «Il 2021 è l'anno peggiore dal 2008: superato il record del 2017». «Incendi: +256% di roghi nell'estate 2021». «Danni per un miliardo». «Andati in fumo 158.000 ettari di bosco». Volutamente, nel ricordare gli articoli, mi sono limitato esclusivamente a quelli che hanno fatto riferimento alle aree, perché non volevo strumentalizzare la sofferenza che abbiamo visto in tantissimi animali, letteralmente bruciati vivi, negli occhi delle persone, vittime, anche loro, della tragedia che ci ha colpito quest'anno, distrutte da questi eventi, messe in ginocchio e in qualche caso addirittura piegate definitivamente, tanto che probabilmente non potranno più riprendersi. Senza considerare la sofferenza di tutti coloro che si sono impegnati attivamente per cercare di limitare i danni di questo dramma. Tutto questo a dimostrazione del fatto che questo provvedimento è non solo opportuno, lecito, legittimo e necessario, ma anche urgente.

è l'emendamento 1.52 (testo 2), che in una discussione così importante, su un tema così rilevante, cerca di introdurre *a latere* il divieto di caccia. Per carità, non sto sindacando sulla sua legittimazione ideologica e non mi sto pronunciando prendendo posizione, perché non è mia volontà farlo ora, ma ritengo sia stato sbagliato introdurre tale tema in questa discussione. So perfettamente che nei dieci minuti che ho a disposizione non potrei convincere nessuno su un tema tanto sentito e radicato nella mente di tutti noi; quindi, non sto parlando del merito, ma del metodo sicuramente, l'opportunità di accelerare l'*iter* approvativo di conversione di un provvedimento così importante, a mio avviso, già da solo avrebbe dovuto escludere la volontà di qualunque intento divisivo di questa maggioranza.

ma di due associazioni che rappresentano centinaia di migliaia di agricoltori, grazie ai quali quotidianamente abbiamo il cibo sulla tavola e grazie ai quali siamo giustamente e legittimamente famosi in tutto il mondo per la qualità delle nostre produzioni: e Coltivatori diretti, che si sono espressi perentoriamente contro questo provvedimento. Lascio a loro il giudizio di merito, ma nel metodo evidenzio di nuovo l'inopportunità di un provvedimento

e dei colleghi del MoVimento 5 Stelle, con l'astensione del Partito Democratico. Quindi, su un provvedimento condiviso al 99 per cento, ritenuto da tutti necessario e non vi è dubbio alcuno sulla necessità di cercare di arrivare alla sua approvazione nel tempo più veloce possibile, si è arrivati ad una votazione di undici-otto a tre. Questo, a mio avviso, dimostra in maniera chiara e inequivocabile quanto poco fosse opportuno cercare di dividere la maggioranza su questo tema. Evidenziata l'unica nota *dolens*, l'unico aspetto per me negativo della discussione attuale, voglio entrare nel merito del provvedimento: un provvedimento - come ho già detto - importante, importante, a mio avviso ben fatto, che però come sempre è migliorabile. Tutto è migliorabile; grazie però alla volontà largamente maggioritaria dell'Assemblea e quindi di tutti i colleghi di arrivare al risultato migliore possibile in parte questo è stato già fatto, grazie ai molti emendamenti presentati, alcuni dei quali a mia prima firma, che hanno ottenuto l'assenso della Commissione, e in altra parte - immagino - verrà fatto dall'Aula. Questo provvedimento, a mio avviso, già nell'articolo 1 contiene un elemento fondamentale: la creazione di una sinergia tra varie forze dello Stato. Oggi è il 26 ottobre e voglio aprire una parentesi che dimostra quanto sia fondamentale

Esercito, Vigili del fuoco, tutti però dipendenti da Ministeri separati. Quindi, per l'Esercito era il Ministero della difesa, per i Vigili del fuoco il Ministero dell'interno, per la Protezione civile la Presidenza del Consiglio dei ministri. Io dicevo, con una battuta, che arrivavano senza nemmeno dire buonasera e cominciavano a fare qualcosa e sono bravi a fare qualcosa - perché era il loro ruolo e venivano mandati per quello. Ma senza un coordinamento succedeva che magari un Corpo perimetrava un edificio che rischiava il crollo e quindi era pericoloso,

necessariamente del buon senso e le persone che operavano in quel momento nel mio Comune il buon senso lo avevano. Quando sono state invitate da me ad un *briefing* pomeridiano - invitate perché io in teoria ero la massima autorità di Protezione civile ma sostanzialmente non avevo autorità nei confronti di nessuno perché, appunto, ero espressione diretta di altri Ministeri - ho spiegato che,

diventando un esempio di gestione dell'emergenza. *(Applausi)*. Dico questo a dimostrazione del fatto che il coordinamento tra le forze dello Stato è indispensabile. Io so - e lo dico per esperienza diretta - che è l'elemento più importante in assoluto nella gestione dell'emergenza,

a quanto previsto nell'articolo 4, comma 2, dove si dice che si finanzieranno gli enti territoriali delle aree interne e, da sindaco di un piccolo Comune della montagna che è anche sede di Parco nazionale, bisogno, quanto sia fondamentale intervenire per la prevenzione in quei Comuni piccoli e montani che non dispongono di risorse proprie, ma rappresentano un'amplissima parte

Quindi è utile e opportuno anche quanto previsto al comma 2 dell'articolo 4, che interviene in queste situazioni di necessità. Ci sarebbe molto altro da dire, ma confido nel fatto che lo faranno i miei colleghi. *(Applausi)*.

Negli ultimi anni abbiamo visto questa emergenza crescere progressivamente e depauperare il nostro territorio del proprio patrimonio forestale e faunistico. Il Sud in particolare, più sottoposto a fenomeni di siccità estrema, ha pagato un caro prezzo in termini di danni ingenti alle proprietà e purtroppo anche in vite umane. È evidente che si tratti di una criticità destinata a crescere per gli effetti del cambiamento climatico e dell'innalzamento progressivo delle temperature medie e massime, come quelle dei fenomeni metereologici estremi, come quelli che si stanno verificando anche in queste ore in Sicilia e in Calabria. Questi eventi hanno ripercussioni che superano il mero impatto immediato sull'ecosistema. I versanti disboscati sono infatti più facilmente sede di fenomeni di erosione accelerata e di frane. I sedimenti che giungono sui fondi vallivi innalzano il proprio alveo, spesso favorendo le alluvioni che possono a loro volta mettere in pericolo vite umane, proprietà, infrastrutture, talora a distanza di chilometri e anche di anni dall'evento. Il decreto-legge al nostro esame affronta alcune delle urgenze e in particolare interviene sul Piano nazionale incendi boschivi per il rafforzamento del coordinamento, l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa sia di previsione che di prevenzione. La Protezione civile è chiamata a valutare e a redigere un *report* con cadenza triennale sulla consistenza ed efficacia dei mezzi e delle azioni realizzate e a considerare eventuali implementazioni. Per far questo si avvale di un comitato tecnico costituito da rappresentanti di diversi Ministeri, della Presidenza del Consiglio dei ministri, che esercita le funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e dei Comuni designati dalla Conferenza unificata. Il comitato per quest'anno ha recentemente adottato un piano, nel quale è riportata una previsione di spesa di 40 milioni, da effettuare entro il 31 dicembre, e comunque complessivamente nel 2021sono investiti in questo provvedimento 150 milioni. È evidente che si tratta di interventi necessari e auspicabili, stante la complessa situazione che si è venuta a creare dopo l'introduzione della legge Madia. Tutti noi dovremmo chiederci se la soppressione del Corpo forestale dello Stato, che doveva garantire risparmi economici ed efficacia degli interventi, ha raggiunto il suo scopo. La cornice legislativa attuale attribuisce le funzioni in materia forestale, ambientale e agroalimentare al Corpo forestale dell'Arma dei carabinieri e la lotta attiva agli incendi al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed è evidente ora il ruolo della Protezione civile, chiamata a svolgere un compito altrettanto importante che in questo caso prevede la gestione tramite un comitato interministeriale a cui intervengono anche le Regioni a Statuto speciale, perché in esse continua a esistere quel Corpo forestale che nelle altre è stato smembrato. C'è, dunque, maggiore efficacia per la filiera decisionale? Sembra che in realtà sia poco efficiente. La riforma Madia ha raggiunto i suoi obiettivi di risparmio economico? Ovviamente no, perché i risparmi annunciati per un triennio erano previsti in circa 125 milioni e noi stiamo stanziando 150 milioni

nel 2018 è passata a 31.700 euro. Inoltre, se si dovessero fare i conti valutando il costo degli interventi demandati ad aziende private in capo alle Regioni, i bilanci sarebbero pesantemente in rosso. Basti pensare che la flotta di Canadair del Corpo forestale dello Stato è stata affidata a società private, che ovviamente badano al loro guadagno, con aumenti esponenziali delle spese.

È evidente la cecità di questa operazione, così come il palese conflitto di interesse di chi lavora per lo spegnimento di un incendio, che teoricamente avrebbe tutto da guadagnare dal fatto che duri più a lungo. Sono aumentate le spese di manutenzione degli elicotteri in dotazione ai Carabinieri; sono aumentati tutti i costi regionali per il contrasto agli incendi boschivi e, malgrado questo, negli ultimi anni si è assistito a un progressivo aumento della durata degli incendi, che comportano danni immani al patrimonio e al contrasto al dissesto idrogeologico. L'aspetto più grave è stato comunque lo spacchettamento delle competenze e la perdita di efficacia,

da assegnare al Ministro dell'interno, per la sua stretta ricaduta in termini di pubblica sicurezza *(Applausi)*. La proposta è di un generale del Corpo forestale dello Stato che conosce bene le criticità e le problematiche di questo settore. Ricordo che le leggi non sono né di Destra né di Sinistra, ma sono utili o meno al Paese e ai cittadini e che il MoVimento 5 Stelle ha sempre messo come priorità i beni comuni e i cittadini. Quale maggior bene comune del bosco? Quale maggiore impatto sulla vita dei cittadini di quello Invito tutti i Gruppi parlamentari ed il Governo a lavorare per soluzioni funzionali sul lungo termine. Con la legge Madia si è data priorità non ai beni comuni, ma alle privatizzazioni e spero sia evidente a tutti il danno che al sistema Paese è stato causato da questo approccio, che alcuni Gruppi politici continuano a perseguire. Si riconoscano gli errori e si pongano rimedi di ampio respiro che guardino al futuro, ad una reale protezione dalle nostre foreste. Questo è quanto fa il MoVimento 5 Stelle.

Signori del Governo, i cambiamenti climatici hanno reso le foreste sempre più esposte al rischio di incendi boschivi. Il migliore strumento di prevenzione degli incendi boschivi è assicurare una gestione sostenibile delle foreste. È assurdo pensare come nel nostro Paese, che ha 11,4 milioni di ettari di bosco, il 38 per cento della superficie nazionale, non si riesca ad attuare un attento monitoraggio ed una corretta pianificazione degli interventi di prevenzione degli incendi boschivi, in base a quanto indicato - peraltro - indicato nella strategia nazionale forestale, la quale, di fronte agli obiettivi perseguiti dal disegno di legge in esame, dovrebbe chiaramente rappresentare un riferimento per mettere in atto le migliori pratiche possibili per il contrasto a tali fenomeni. Anche questo è stato più volte segnalato dall'UNCEM. In tal senso, esprimiamo comunque soddisfazione alla Commissione ambiente per l'approvazione dell'emendamento 5.23, con il quale si prevede che le attività di prevenzione selvicolturale degli incendi boschivi e la programmazione dei fondi strutturali siano collegate alle migliori previsioni sull'evoluzione delle compagini forestali, contenute negli innovativi strumenti di pianificazione forestale previsti dall'articolo 6 del testo unico delle foreste, con particolare riguardo alla strategia forestale nazionale, tema importantissimo. Lo scorso 16 luglio la Commissione europea approvato la nuova strategia per le foreste per il 2030. Se si confrontano gli obiettivi europei con i contenuti della strategia nazionale, si possono individuare le azioni prioritarie di intervento, per raggiungere risultati soddisfacenti in tema di prevenzione e soprattutto e soprattutto di sostenibilità. In base agli studi, se da un lato infatti l'Italia rivela buone prestazioni per le misure di tutela ambientale di tipo passivo, dall'altro appare assolutamente in ritardo sui sistemi di monitoraggio e di pianificazione, cioè sulle misure di tipo attivo. È su questo tema che dobbiamo lavorare. I dati dimostrano che il primo fattore predisponente per un incendio è dato dalle condizioni meteorologiche e climatiche: la siccità, l'aridità, le alte temperature, la bassa umidità, la forte ventosità, l'alta frequenza di eventi estremi, quali le ondate di calore, sono i fattori in in presenza dei quali un incendio può facilmente acquisire vigore ed interessare vastissime superfici. In questa prospettiva è fondamentale tornare a valorizzare le modalità organizzative del settore forestale italiano, così da raggiungere un livello ottimale di monitoraggio del territorio e prevenzione di questi fenomeni. Tale prevenzione trova nella gestione forestale sostenibile, con riguardo anche al potenziamento della viabilità forestale questo è un nostro emendamento, il 4.22 - e quindi anche nell'attivazione di misure per la pianificazione, il superamento della frammentazione fondiaria, la creazione di filiere economiche e la valorizzazione dei servizi ecosistemici ambientali forniti dal bosco e i suoi fondamentali. È questa la gestione forestale che deve essere promossa, al fine di avere strumenti di gestione efficaci per il futuro. In tal senso, un tema importante che deve essere immediatamente affrontato è la scarsità di risorse economiche di cui dispone la strategia forestale nazionale. In questa direzione, ricordo a questa Assemblea che si era mosso il primo Governo della Lega di questa legislatura, con il ministro Centinaio *(Applausi)* che a guida del Ministero delle politiche agricole e forestali, con la legge di bilancio del 2019, ha istituito il fondo per le foreste italiane, con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per il 2019,

È necessario, dunque, individuare fin da subito gli strumenti di natura finanziaria volti a incrementare l'attuale disponibilità di questo fondo per un'efficace azione di cura e gestione di questo importantissimo patrimonio verde, che oggi è in continua espansione, ma anche in un lento stato di abbandono. Una risorsa abbandonata è una risorsa per la quale non viene riconosciuto un valore e che per questa ragione non viene monitorata. La prevenzione a costi minori è quella connessa alla rivitalizzazione dell'economia del settore. Un bosco che produce valore, legname, biomassa, funghi, tartufi, castagne, ma anche servizi turistici, ricreativi, culturali è un bosco che viene difeso e, quindi, difficilmente brucia.

L'emendamento 1.44 (testo 2), che è stato ripresentato in questa fase, è importantissimo perché dà all'agricoltore la possibilità di svolgere questo ruolo.

Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, siamo qui per convertire in legge un decreto-legge varato lo scorso settembre per far fronte all'emergenza dovuta ai numerosi e drammatici incendi che hanno interessato nel corso dell'estate il nostro Paese e, in particolare, la mia Regione, la Calabria. L'*escalation* di fuoco ha toccato tutta l'Italia per un totale di 140.000 ettari di boschi bruciati solo nel 2021. Tale dato è stato riportato ampiamente dalla stampa. In Calabria i danni maggiori alle aree forestali si sono verificati nel Parco nazionale dell'Aspromonte, dove sono andate distrutte aree di bosco secolare, una perdita di patrimonio inestimabile.

Mentre si cerca di puntare il dito su presunti piromani seriali, che esistono, anche se in misura residuale, si distrae lo sguardo dagli interessi che spesso sottendono tali atti criminosi. dagli incendi per creare nuovi pascoli a quelli appiccati per saccheggiare ciò che è sopravvissuto alle fiamme a scopo di lucro, fino al *business* legato ai rimboschimenti e relativi finanziamenti. questo decreto incendi, nonostante contenga delle buone misure ridisegnando la *governance* della prevenzione incendi e stanziando le risorse per potenziare la capacità operativa delle componenti statali impegnate nella lotta ai roghi, non risolve, a mio modesto avviso, il problema degli incendi

Bisognava agire, a mio modesto avviso, su più fronti. A questo proposito ho presentato anche io diverse proposte emendative che, in sede di trattazione in Commissione, non sono state tutte accolte, anche se alcune lo sono state in parte. di primaria importanza era e sarà in futuro l'introduzione di alcuni divieti perenni e non più limitati a un periodo di tempo riguardanti le zone percorse dal fuoco. Uno degli emendamenti stabiliva il divieto perenne di prevedere una destinazione diversa da quella che dette zone avevano prima dell'incendio. In questo modo si sarebbe evitato ogni possibile rischio di incendio di origine dolosa messo in atto al fine di poter utilizzare successivamente le aree boscate distrutte dal fuoco a vantaggio di interessi privati, seppur dopo alcuni anni. Molto spesso bruciare equivale a costruire in un momento successivo (per questo, secondo me, il divieto perenne era e sarà importante), considerando il bosco come un bene economico da sfruttare per interessi meramente privatistici. L'emendamento nella nuova formulazione è stato completamente stravolto, perché non va a toccare - come da me proposto - il comma 1 dell'articolo 10 della famosa legge n. 253 del 2000, relativo ai divieti anzidetti, ma il comma 2, precisando che anche la superficie percorsa da controfuoco la superficie percorsa da controfuoco rientra nel perimetro finale dell'incendio, con tutte le conseguenze del caso. Questa è comunque una cosa buona, ma la portata di tale modifica è marginale rispetto a quanto avevo originariamente proposto, dopo aver interloquito con Federparchi e con tantissimi enti *no profit* che hanno a cuore il bosco. Lo stesso dicasi per un'altra mia proposta che stabiliva che stabiliva la mancata corresponsione delle risorse ai Comuni che non approvino gli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco entro i limiti fissati dalla legge. In questa nuova formulazione, che anche parzialmente stravolge il mio emendamento, alle Regioni il potere sanzionatorio sui Comuni inadempienti. Penso alla mia Regione: essa stessa è stata spesso - troppe volte, in passato - inadempiente. Quindi mi pare che si passi dalla padella alla brace. Penso alla mia Regione, alla Calabria, e tutto questo da parlamentare mi fa riflettere. Ecco perché questa misura non servirà, secondo me, a garantire il tempestivo aggiornamento degli elenchi dei soprassuoli. Spero di sbagliarmi. Son contento però che la Commissione abbia approvato l'emendamento a mia prima firma che prevede che facciano parte del comitato tecnico - come da me proposto - anche qualificati rappresentanti delle associazioni di volontariato iscritte nel nuovo registro unico nazionale del terzo settore e impegnate nella lotta agli incendi boschivi. Questa è una cosa molto bella e importantissima. Ciò consentirà al comitato di assumere un punto di vista importante per analizzare i rischi e stabilire le politiche di prevenzione (la prevenzione appunto, tanto importante) e di lotta agli incendi, soprattutto ai fini della redazione del Piano nazionale. Tuttavia ho qualche perplessità, perché nella riformulazione sono state aggiunte anche le associazioni con finalità di protezione degli animali e dell'ambiente e le organizzazioni di rappresentanza delle imprese agricole. Qui perdonatemi - ho colto con più difficoltà il senso di questa riformulazione. Uno degli emendamenti a mia prima firma prevedeva peraltro anche la modifica di una norma contenuta nella legge di bilancio del 2020 (legge n. 178), la quale prevede che l'assunzione di questi lavoratori, che oggi sono a tempo determinato (come la suddetta prevede, con scadenza

anche solo immaginabile, tra gli incendi e qualunque provvedimento di proroga di rapporti di lavoro a tempo determinato. Lo ripeto: si sarebbe dovuto evitare ogni nesso di causalità fra gli incendi e qualunque provvedimento di proroga di rapporti di lavoro di lavoro a tempo determinato. Questo è stato anche oggetto di tante riflessioni con i parchi, i presidenti e gli enti *no profit*. Occorreva stabilizzare i lavoratori; chi mi conosce sa quanto ho fatto in questi anni, in Governi diversi, per stabilizzare altre platee. Continuerò a portare avanti questa battaglia a tutela non solo dei lavoratori precari e a tempo determinato, ma anche del bosco. Di fondamentale importanza era altresì, secondo me, approvare la modifica riguardante la flotta dei Canadair - un collega ne ha parlato poco fa contenuta in un altro emendamento. La mia proposta prevedeva di abolire i contratti di esercenza della flotta Canadair stipulati dal Dipartimento dei vigili del fuoco con società private e di reclutare invece i piloti nel corpo dell'Aeronautica militare. In questo modo, si sarebbe evitato ogni probabile rischio di interessi privatistici nella lotta agli incendi e quindi quindi avremmo fatto i conti con un notevole risparmio di soldi pubblici. Secondo i dati riportati dalla stampa, l'appalto dei Canadair ha un costo di 360 milioni di euro, a cui vanno ad aggiungersi le ore di volo in più rispetto a quelle previste dalla gara (3.500 all'anno). Il costo di un'ora di volo

estera che, dal 15 giugno al 22 settembre 2021, ha effettuato 5.147 ore di volo. Conti alla mano, converrebbe indubbiamente formare i piloti e optare per la gestione pubblica. Questo è un suggerimento che rivolgo al Governo. Non mi dilungo Non mi dilungo oltre. La prevenzione è la cosa che mi sta più a cuore ed è la parola d'ordine per proteggere i boschi, che sono ecosistemi senza i quali qualsiasi tentativo di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici risulterà vano. È fondamentale comprenderne a fondo l'enorme valore per i territori. Spesso gli effetti

al potenziamento della prevenzione degli incendi e a scongiurare ogni possibile rischio di comportamenti dolosi. Mi auguro che tutto questo possa essere approvato in successivi emendamenti e provvedimenti. *(Applausi)*.

va detto subito che il decreto-legge in esame è quanto mai attuale. La Sardegna sta bruciando ancora, anche in queste ore, segno che il tempo metereologico favorevole, tuttora caldo e asciutto, la espone al rischio di incendi dall'inizio dell'estate fino all'autunno inoltrato. Proprio nella giornata di sabato scorso, 23 ottobre, si sono registrati ben dieci incendi sul territorio regionale. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale ha autorizzato anche i mezzi aerei del sistema regionale antincendio, oltre a mettere in campo squadre a terra.

Per diversi giorni e notti in Sardegna sono andati avanti roghi divampati su più fronti nei boschi del Montiferru e nelle campagne attorno al Monte come ampiamente trasmesso dalle televisioni locali e nazionali. Il bilancio è stato di più di 1.000 persone costrette, insieme agli ospiti di un'intera casa di riposo, a lasciare le loro abitazioni e, alla fine della conta, di circa 12.000 ettari di bosco (tra cui olivi millenari, pascoli e macchia mediterranea) andati in fumo, senza parlare della morte di molti capi di bestiame, bruciati o soffocati.

Negli stessi giorni, un altro incendio ha devastato 1.500 ettari, di cui 400 boschivi, nella zona del Monte Arci, sempre in Sardegna. Sono notizie che noi sardi non vorremmo mai leggere, tanto vasti sono il danno e la disperazione che ne è seguita. decreto-legge è stato adottato i primi di settembre, dopo che anche altri territori d'Italia avevano preso fuoco. Si sono riscontrate ovunque difficoltà a contenere gli incendi e si è preso amaramente atto che il dispositivo andava rinforzato. È evidente che il pregio di alcune zone d'Italia è quello di avere ampie superfici boschive e una natura largamente preservata, ma questo, che è un evidente valore, può rappresentare anche una fragilità.

La Sardegna, in particolare, è considerata un'oasi tanto bella, quanto fragile e delicata, con una superficie boscata amplissima, ma difficile da controllare, stante il territorio largamente montuoso e collinare. Nell'isola si aggiunge il problema della discontinuità territoriale, un tema che affronteremo a breve nel disegno di legge costituzionale. Gli incendi a ridosso dei confini tra Regioni limitrofe si possono infatti estinguere anche usando le squadre di spegnimento di più Regioni, ma in Sardegna no. Rafforzare quindi le squadre di spegnimento aereo anche a livello centrale può essere utile per raggiungere pure i luoghi più isolati; in Sardegna, ad esempio, quest'estate sono arrivati persino due Canadair dalla Francia e dalla Grecia, ricorrendo al meccanismo europeo di protezione civile: per fortuna che esiste, in questo caso, anche l'Europa solidale rispetto alle chiamate della

Le norme vanno non solo a integrare quelle esistenti, ma puntano proprio a ottimizzare il dispositivo operativo. Potremmo definirlo un vero e proprio piano di lotta contro gli incendi boschivi. Che cosa serve ora per scongiurare episodi gravi come quelli nelle zone del Montiferru? Bisogna lavorare ancora sulla previsione, cioè capire quando determinate aree a causa delle condizioni metereologiche diventano sensibili agli incendi, e quindi bisogna agire sulla prevenzione dei roghi, che nella maggior parte dei casi sono originati, spesso con dolo, proprio dall'uomo. È pertanto fondamentale avere mezzi e uomini, ma soprattutto una serie di strumenti in grado di favorire un coordinamento ancora più efficiente tra chi opera sul campo, i corpi dello Stato e tutti gli enti del territorio. Le azioni per contenere gli incendi e limitare i danni, che spesso si verificano nei medesimi periodi, richiedono l'intervento di più uomini e mezzi aerei e terrestri, ed è quindi quanto mai opportuno affidare al Dipartimento della protezione civile, che forse è stato un po' troppo spezzettato negli anni, la ricognizione e la valutazione degli strumenti innovativi. Ormai non si può più lasciare solo alle vedette - che sono importantissime, dove ci sono - l'avvistamento dei focolai; ci sono tecnologie sempre più sofisticate, anche satellitari, che devono andare a integrare i sistemi di previsione, sorveglianza, monitoraggio e rilevamento dell'ambiente. Per gli uomini che operano nello spegnimento degli incendi servono sia i mezzi sia una formazione ulteriore. Serve inoltre un maggiore e migliore coordinamento tra i piani antincendio regionali e quello nazionale. I piani regionali devono: puntare soprattutto sulla prevenzione; contrastare l'abbandono di attività di cura del bosco; prevedere postazioni di atterraggio dei mezzi di soccorso; realizzare infrastrutture come, ad esempio, nuove vasche di rifornimento idrico utili per accelerare gli interventi di spegnimento di incendi; predisporre vie d'accesso e tracciati spartifuoco e la manutenzione delle aree periurbane. Insomma, è necessario un potenziamento della risposta al fenomeno degli incendi boschivi, migliorando la capacità operativa di chi deve coordinare gli interventi e di chi li deve realizzare sul campo. Servono anche disposizioni che potenzino, da un punto di vista giuridico, la prevenzione e la repressione degli incendi, attraverso una revisione e un'integrazione delle prescrizioni in materia di obblighi, divieti e sanzioni. Occorre quindi non solo l'inasprimento delle sanzioni, ma anche la necessità di colpire gli interessi degli autori degli illeciti, incentivando la collaborazione con le indagini e favorendo le condotte volte alla riparazione del danno causato. Spesso, a causare gli incendi nei boschi è chi dovrebbe tutelarli, quindi ci pare opportuno prevedere aggravanti per questi casi e attenuanti per chi voglia invece riparare il danneggiamento. A noi sembra che il decreto-legge in esame vada proprio nella direzione giusta.

Cosa faranno queste persone nel frattempo? Staranno a guardare l'erba che cresce, senza poterla utilizzare per i loro animali?

come potranno essere utilizzate da parte degli abitanti? È questo il problema che sottopongo a voi, onorevoli membri del Governo. Esistono disposizioni

Altri colleghi hanno fatto presente la necessità di perimetrare in misura ancora maggiore le aree che purtroppo sono state oggetto di questi eventi devastanti, che hanno colpito la natura in maniera drastica. Orbene,

una perdita di tempo talmente grande che, quando la legge verrà pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, chi dovrà beneficiarne dovrà andare a guardare per capire esattamente quale parte può usare e quale no, non considerando le Regioni, su cui piomberà addosso

a cinque anni dalla sua entrata in vigore, oggi possiamo dire con certezza che la legge Madia, approvata durante il fallimentare Governo Renzi, è stata un clamoroso disastro, e andiamo a spiegare il perché. Ricordate il Corpo forestale dello Stato? Immagino di sì, anche perché esisteva dal 1822, quasi duecento anni di onorato servizio, finché non è arrivato al Governo chi decise di decapitare cotanta storia e competenza al servizio delle persone e dell'ambiente (era il 2016).

alcuni miseri milioni di euro; pochi, pochissimi, miserabili milioni di euro per sacrificare un corpo specializzato che salvava vite, umane e animali, e l'ambiente dagli incendi, con competenza e coraggio, presente soprattutto a terra, perché gli incendi si spengono a terra, col paradosso poi - non possiamo dimenticarlo - che, a fronte dello scioglimento del Corpo forestale dello Stato, sono rimasti in vita cinque corpi forestali delle Regioni a Statuto speciale. Abbiamo quindi un'Italia a macchia di leopardo in materia di antincendio boschivo, dove di fatto tutto o quasi è bloccato a causa della mancanza di coordinamento tra le forze interessate alla prevenzione e allo spegnimento degli incendi; dove migliaia di operatori forestali presenti sul territorio sono stati fatti confluire in talmente tante altre diverse amministrazioni pubbliche da perderne il conto: Carabinieri, Vigili del fuoco, Polizia dello Stato, Guardia di finanza e Ministero delle politiche agricole, Tale frantumazione delle competenze ha portato a un sostanziale abbandono del territorio, senza dimenticare la miserabile fine che ha fatto la flotta di elicotteri antincendio in dotazione al Corpo forestale, forestale, che è stata smembrata e smantellata, proprio come i suoi piloti, che oggi non volano più, e che ha costretto lo Stato a fare affidamento ai privati, con un aggravio dei costi che urla vendetta: si parla - udite bene! - di più di 15.000 euro pagati ai privati per ogni ora di utilizzo dei Canadair per spegnere le fiamme, quando prima queste operazioni venivano eseguite dai piloti e dagli elicotteri del Corpo forestale dello Stato, con costi infinitamente inferiori. Oggi questo disastro è sotto gli occhi di tutti, con migliaia di incendi devastanti, che hanno percorso i nostri boschi, uccidendo persone, animali selvatici e ambiente, e con danni miliardari, a fronte di un risparmio di soli 30 milioni di nel triennio 2017-2019, come ha rilevato recentemente la Corte dei conti. Si tratta di un risparmio che ovviamente non esiste, se valutiamo i maggiori, ingentissimi costi conseguenti all'aumento degli ettari di terreno andati in fumo. Per capire, solo per i roghi del 2021, quindi di questi mesi, si parla di danni per almeno un miliardo di euro: non so se ci rendiamo conto di ciò che è accaduto. forse, nessuno - ne parlano. O meglio, si parla e si è parlato degli incendi e dei danni che provocano, ma lo si fa come se si parlasse di eventi inevitabili, a cui ci dovremmo abituare. Invece, si sarebbero potuti limitare e questo bisogna dirlo a gran voce agli italiani. I maggiori danni provocati dagli incendi di quest'ultimo periodo sono anche la conseguenza dei ritardi negli interventi per lo spegnimento. Questi ritardi dipendono dall'eccessiva burocrazia, con conflitti di competenze tra le diverse amministrazioni, e da una generale mancanza di coordinamento. *(Applausi)*. Dobbiamo avere il coraggio di dire che erano incendi che si sarebbero potuti spegnere in meno tempo e quindi con meno danni. Sarebbe stata sufficiente la presenza di una polizia forestale e ambientale ben radicata sul territorio, esattamente come lo era il Corpo forestale dello Stato. Un dato su tutti è sconcertante:

su tanti ambiti già da molti anni, ad esempio aumentando esponenzialmente le risorse destinate al Corpo forestale dello Stato e non cancellandolo, come ha fatto il Governo Renzi, con la cosiddetta riforma Madia, nel 2016. Tutte le forze politiche oggi devono lavorare concretamente per l'ambiente e contrastare attivamente il cambiamento climatico, seguendo l'unica via possibile, che è quella della transizione ecologica. Citiamo qualche dato ulteriore: fino al 31 dicembre 2016, il perno del sistema di coordinamento esistente in materia di antincendio boschivo era il Corpo forestale dello Stato. Lo dico piano: fino ad allora,

che è stato scritto appunto per cercare di "mettere una pezza" al caos. È difficilissimo mettere una pezza a un abito che non può più essere assolutamente rammendato, ma si cerca di creare un miglior coordinamento tra tutte le forze interessate allo spegnimento degli incendi. Abbiamo visto infatti che tali forze sono divise tra tante, diverse amministrazioni, che si accavallano, bloccando e abbandonando il territorio. Dobbiamo anche essere onesti nel dire che questo decreto-legge, seppur cerca di intervenire, non può bastare a evitare che nei prossimi anni centinaia di migliaia di ettari

sul territorio, vicino ai luoghi degli incendi, e in grado di intervenire immediatamente. L'unica strada è questa, oltre alla lotta al cambiamento climatico.

soprattutto che l'unica soluzione è una nuova polizia civile forestale e ambientale. Non c'è più tempo da perdere: ricreare un corpo civile specializzato è l'unica soluzione; se non la intraprendiamo il prima possibile, un giorno ci troveremo a dire che è troppo tardi, anche perché non c'è altro destino che questo. Bisogna solo decidere quando farlo e, se non sarà subito, come chiede il MoVimento 5 Stelle, vorrà dire che saremo destinati a contare ogni estate i danni che avremmo potuto evitare, e ciò non è accettabile. Chiediamo pertanto a tutte le forze politiche interessate di appoggiare queste iniziative e anche al presidente Draghi di prendere una posizione netta, che garantisca l'appoggio del Governo sul ritorno della polizia forestale civile. Il tempo, signor Presidente, è finito e la nostra bellissima Italia, con la sua meravigliosa e unica biodiversità, non può più aspettare. *(Applausi)*.

che sicuramente offrirà una risposta migliore rispetto a quella data fino a oggi dalla nostra legislazione, ma naturalmente ancora tanto bisogna fare e prevedere, soprattutto in una logica che non sia sempre quella della decretazione di urgenza. Colleghi, sapete tutti che questa è stata la peggiore stagione degli incendi in Italia da trent'anni a questa parte: il 12 per cento del patrimonio forestale nazionale e sono 150.000 gli ettari di bosco andati a fuoco in Italia dall'inizio dell'anno. Trent'anni sono tantissimi. Se ognuna delle persone che hanno parlato degli incendi e se ognuno dei passati Governi che hanno scritto su questa materia

Non tutti sanno che il patrimonio forestale italiano è tra i più importanti d'Europa per ampiezza e varietà di specie e costituisce un'immensa ricchezza per l'ambiente e l'economia, per l'equilibrio del territorio, per la conservazione della biodiversità e del paesaggio. Il nostro è veramente il più importante d'Europa, quindi è un costo drammatico quello che l'Italia è stata costretta ad affrontare, perché è mancata l'opera di prevenzione nei boschi, che, a causa dell'incuria e dell'abbandono, sono diventate vere giungle ingovernabili. Abbiamo assistito inerti all'inarrestabile avanzata della foresta, che senza alcun controllo si è impossessata di territori incolti e domina ormai più di un terzo della superficie nazionale, con una densità che la rende del tutto impenetrabile ai necessari interventi di manutenzione, difesa e sorveglianza. Voglio però evidenziare, colleghi, che dall'Unità d'Italia questa superficie è raddoppiata e oggi copre 11 milioni di ettari. Da siciliana, la prima cosa che mi viene in mente è che tutti questi terreni, in effetti, sono rimasti abbandonati. Come diceva anche il collega Floris, le aziende agricole man mano scompaiono, per dieci anni vengono penalizzate e paralizzate

contrastino l'allontanamento dalle campagne, perché si possano appunto valorizzare le funzioni di sorveglianza, manutenzione e gestione del territorio svolte proprio dagli imprenditori agricoli, dai nostri imprenditori agricoli.

dei nostri *social media* per farci rendere conto di quello che stava succedendo. Abbiamo incendi molto più rapidi, intensi e di larghe dimensioni;

la colpa, che invece è dei comportamenti dolosi di una moltitudine di soggetti, come pastori in cerca di pascoli più ricchi e puliti, incendiari con motivazioni vendicative, operai forestali in cerca di future opportunità di impiego, cacciatori interessati a controllare e concentrare le aree di rifugio della selvaggina o raccoglitori di prodotti selvatici. La causa prevalente degli incendi però sono i comportamenti colposi, collegati a noncuranza, negligenza, imperizia e sottovalutazione del rischio. Nell'Europa meridionale, il 70 per cento degli incendi è legato proprio

di prevenzione, che, da una parte, viene definita indiretta, cioè legata alle pratiche colturali che permettono la scelta di specie appropriate e la realizzazione di diradamenti e di interventi di pulizia del sottobosco, sottobosco, che hanno un'importanza fondamentale per aumentare la resistenza e la resilienza delle formazioni forestali. Abbiamo poi anche una prevenzione diretta, che significa - come hanno detto i miei colleghi - realizzazione e manutenzione di fasce tagliafuoco, riduzione del materiale combustibile e pulizia delle fasce laterali,

le differenze in termini di investimento economico delle due opzioni, perché la prima interessa i piccoli operatori del mondo rurale, mentre la seconda, quella dello spegnimento, coinvolge soggetti esterni del settore forestale, in particolari aree del *business* connesse alla flotta connesse alla flotta aerea e ai sistemi di monitoraggio, settori formalmente legati all'industria militare. Della foresta abbandonata abbiamo parlato tutti, ma voglio richiamare solo un dato che vorrei fosse valutato attentamente: se, da una parte, vietare per proteggere e ricostruire il patrimonio va bene, dall'altra però ritengo, soprattutto da donna a una forza politica in cui si privilegiano il lavoro, il reddito e l'imprenditoria, che gestire il patrimonio e valorizzarlo anche economicamente per ridurre i costi della sua tutela sia molto meglio. È una cultura, questa, che purtroppo abbiamo ereditato dalla fine dell'Ottocento, quando il Paese si era dotato di una rigida normativa di vincolo dei territori boscati e di una Forza di polizia specializzata nella tutela delle risorse forestali. Questa superficie in cinquant'anni si è raddoppiata e vale quindi la pena di di trovare formule per cui il costo di una gestione, dando una valorizzazione alle foreste, sarebbe sicuramente minore a quello della prevenzione. Poi abbiamo un problema di *governance,* che ha ampiamente documentato il collega Toninelli

Il provvedimento affida al Dipartimento di protezione civile il compito di affrontare, con cadenza triennale, il Piano nazionale per il rafforzamento delle risorse umane, tecnologiche, aeree e terrestri necessarie per prevenire e contrastare gli incendi boschivi; documento che andrà a integrare la consueta pianificazione regionale. Spero che il coordinamento strutturato con l'apparato centrale dello Stato possa finalmente garantire maggiori risorse alle Regioni per combattere questa piaga. Tra le novità più rilevanti che spero possano trovare piena e rapida applicazione, vi è la ricognizione e valutazione, che viene affidata al Dipartimento della protezione civile, di strumenti innovativi, con le nuove tecnologie che oggi possono sicuramente dare un grande aiuto. Penso a quella satellitare, idonea all'integrazione di sistemi di sorveglianza, monitoraggio e rilevamento dell'ambiente, ai droni, al controllo remoto, mezzi capaci di rilevare in tempi rapidissimi anche piccoli focolai di incendio. I mezzi messi a nostra disposizione dalla tecnologia aerospaziale sono oggi straordinari. Se venissero sfruttati appieno e ben coordinati, la battaglia contro il fuoco

devo dire che il provvedimento di cui stiamo trattando ha un'importanza particolare, perché dopo l'estate del 2021, che è stata particolarmente particolarmente complicata dal punto di vista della lotta agli incendi, credo si sia acquisita anche una necessaria consapevolezza di quanto questo cancro, che va a colpire il nostro patrimonio forestale debba essere debellato con ogni sforzo. Lascerei perdere in questo senso alcune, diciamo, suggestioni climatiche come quelle che ci ha riportato prima il senatore Toninelli, che certamente avranno la loro ragion d'essere in qualche altro luogo del mondo, ma che temo poco abbiano a che fare con incendi dolosi appiccati essenzialmente nel Sud Italia e in alcune zone ben specifiche. Ecco, interroghiamoci a partire da questo: come mai in alcune aree del Paese si sviluppano così facilmente incendi e come mai combattere in quei territori il fuoco all'interno delle aree boscate è sempre un'impresa titanica. A fronte di questo, bisogna prendere consapevolezza che il quadro penale, come è stato affrontato anche in questo provvedimento, necessita di essere messo a fuoco. Sono necessarie azioni di contrasto alla criminalità che si nasconde dietro agli incendi boschivi. Non raccontiamoci che i fuochi si sviluppano da soli, perché tale fenomeno in natura è cosa estremamente rara e certamente totalmente avulsa dal contesto di cui stiamo parlando. Parliamo invece degli interessi che stanno dietro a chi incendia boschi, non solo degli interessi legati a chi, magari prima della stessa legge del 2000 che impedisce il cambio di destinazione d'uso del territorio, pensa di utilizzare questo strumento appunto per modificarne la destinazione d'uso, come avveniva molti anni fa.

come quello di chi combatte gli incendi o la Protezione civile o altri, dobbiamo essere molto determinati e addirittura - come è il caso - se qualcuno viene trovato a commettere questo tipo di reati, colpirlo gravemente Bisogna avere il coraggio di affrontare questi tabù, altrimenti c'è sempre l'idea di una manina nascosta, che non si sa a chi appartenga, che va ad accendere i fuochi. Magari bisogna

impedendo che ci sia un vuoto all'interno degli organici dei Vigili del fuoco, soprattutto per quanto riguarda il *turnover.* Inoltre occorre anche mettere mano, in maniera

in qualche caso anche di ambiguità tra chi l'incendio lo deve spegnere e chi purtroppo, come abbiamo visto in qualche indagine del mese di agosto di quest'anno, l'incendio lo appicca. Vedremo come si sviluppa anche il resto delle votazioni, perché riproporremo in Aula delle opportunità per il Governo di prendere posizione. Anche in questo senso mi spiace che il Sottosegretario si stia allontanando dall'Aula; evidentemente non ha interesse per l'argomento. Detto questo, andiamo avanti in maniera determinata. Abbiamo inserito nel provvedimento la riduzione a cinque mesi

con tempi più abbreviati e quindi riducendo l'accumulo di ritardo che si è verificato a partire dal tempo del Covid.

Vedremo poi se all'interno della legge di bilancio saranno ricompresi - ne siamo certi - i provvedimenti che riguardano lo sgravio dei costi dell'IVA per i volontari per l'acquisto dei mezzi antincendio e delle attrezzature. Abbiamo raccolto con molta soddisfazione il favore del Governo; ovviamente si tratterà di passare dalle parole ai fatti, essendo chiaro che nel provvedimento in discussione la capienza economica era ridotta. Auspico tuttavia che il rinvio alla legge di bilancio sia solo questione di tempo e non di mancanza di volontà. Come ho già detto occorre la consapevolezza che il nostro Paese è troppo spesso sulle cronache per problemi legati agli incendi,

in maniera determinata in questo sforzo; se si tratta di combattere la criminalità che sta dietro a chi appicca gli incendi, dobbiamo essere tutti uniti in questo sforzo e l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno è che su un provvedimento così importante si inseriscano divisioni ideologiche su basi che nulla c'entrano con la lotta agli incendi, come stavamo dicendo a proposito

il ministro Costa, che veniva dal Corpo forestale dello Stato: è al Governo da più o meno a tre anni e mezzo e se avesse avuto veramente la volontà di ricostituire il Corpo forestale dello Stato, aveva tutte le opportunità, quando era Ministro del Governo ed anche in questi anni per poterlo fare. Evidentemente, è più utile venire in Aula e fare dichiarazioni di principio che mettersi poi di impegno seriamente e fare le cose. *(Applausi)*. Un ringraziamento va ai nostri Vigili del fuoco e ai volontari della Protezione civile, che si battono costantemente nelle situazioni di incendio, di pericolo, che mettono a rischio la vita stessa delle persone. Dobbiamo dare a costoro non solo la certezza che lo Stato mette a disposizione gli strumenti materiali per spegnere gli incendi, ma anche le risorse umane per non essere pochi

ma occorre necessariamente anche rimpinguare, come anche le forze sindacali stanno a gran voce chiedendo al Governo, con assunzioni straordinarie gli organici dei Vigili del fuoco. Solo con un dispositivo ben distribuito sul territorio potremo essere all'altezza di combattere operativamente ogni forma di incendio.

Signor Presidente, come detto, il provvedimento che ci accingiamo a votare pone l'attenzione su un fenomeno criminale che sta minando gli ecosistemi, la sicurezza dei territori e la loro tenuta idrogeologica, oltre che attentare alla vita di persone e animali. Un suolo percorso dal fuoco perde valore, generando conseguenze nefaste anche sull'economia e mettendo spesso in crisi le aziende, gli imprenditori e le loro famiglie. La cronaca della scorsa estate ci ha quotidianamente informato sull'enorme numero di incendi, i dati dello European Forest Fire Information Systems riportano un quadro disarmante: sono stati bruciati oltre 158.000 ettari di aree boscate, di macchia e agricole, pari alle superfici dei territori comunali di Roma, Milano e Napoli. Una tragedia che ha interessato in modo particolare tre Regioni, Sicilia, Calabria e Sardegna, senza che l'azione incendiaria risparmiasse Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Abruzzo. Secondo la Coldiretti, serviranno almeno quindici anni per ricreare il patrimonio verde cancellato dalle stesse fiamme che hanno distrutto pascoli, coltivazioni, fienili e mezzi agricoli, ma anche ucciso un numero non quantificabile di animali da allevamento e selvatici, questi ultimi patrimonio dello Stato e di biodiversità. Il Ministero dell'interno nell'arco della scorsa estate ha registrato circa 80.000 interventi di spegnimento o contenimento, in forte aumento rispetto all'anno precedente, con quasi 25.000 operazioni in più. Inoltre, gli incendi nelle aree protette sono stati 756 nei parchi nazionali e 1.310 nei parchi regionali. È una situazione drammatica per l'intero patrimonio naturale. L'uomo è la principale causa di questo scempio. A sottolinearlo è il WWF, secondo il quale il 96 per cento degli incendi sono legati alle attività antropiche; spesso gli atti dolosi sono espressioni di interessi speculativi legati ai servizi antincendio o al mercato fondiario. A questi si aggiungono gli incidenti derivanti da negligenza, da cause accidentali o da cattive pratiche agronomiche come l'insensata abitudine, ancora troppo diffusa, di pulire i terreni agricoli bruciando i residui vegetali e finendo per distruggere materia organica che viene così sottratta alle colture. Non dobbiamo commettere, però, l'errore di associare tra loro le molteplici cause degli incendi appiccati per motivi diversi concorrendo a ciò che solo apparentemente si mostra come un disegno unico. Alla luce delle cause citate e delle difficoltà che ogni anno l'Italia affronta nel tentativo di ridurre i danni procurati dagli incendi, la prevenzione assume un ruolo di primo piano. Gravissima è la stima fatta da Europa Verde, secondo la quale il 44 per cento dei Comuni italiani non ha attivato il catasto incendi, fondamentale per segnalare le aree percorse da fuoco e vincolarle per i successivi anni, al fine di contrastare la speculazione edilizia, agricola e pastorale. Anche laddove attivato, non sempre gli enti preposti forniscono i dati planimetrici e li trasmettono ai Comuni, rendendo inefficace questo strumento. Neanche l'attività normativa posta in essere negli ultimi anni ha migliorato la situazione. Il decreto legislativo n. 177 del 2016, la cosiddetta riforma Madia, ha cancellato il Corpo forestale dello Stato, specializzato nella tutela tutela dell'ambiente e dell'agroalimentare nazionale, portando alla militarizzazione forzata di 7.000 dipendenti civili, penalizzando la tutela del patrimonio boschivo e le operazioni antincendio, senza portare alcun effettivo risparmio alle casse dello Stato, come spiegava bene il collega Toninelli. Oggi abbiamo l'obbligo di ripensare il sistema di prevenzione degli incendi aumentando le risorse finanziarie per potenziare le capacità operative con specifiche previsioni a favore delle strutture dedicate nelle isole minori e nelle aree interne in cui il rischio di incendio è elevato. molto positivi i contenuti del provvedimento in discussione come, ad esempio, il potere sostitutivo delle Regioni nel caso in cui i Comuni non provvedano ad aggiornare il catasto incendi e la redazione da parte della Protezione civile di un Piano nazionale triennale di aggiornamento tecnologico delle azioni di prevenzione e lotta attiva agli incendi, cui sono dedicate specifiche risorse per acquistare nuovi mezzi operativi fondamentali nelle operazioni di spegnimento. Vengono anche inasprite le pene per gli incendiari, deterrente necessario per la prevenzione. Viene, inoltre, stanziata la somma di 100 milioni di euro in favore degli enti territoriali per interventi volti a prevenire gli incendi boschivi nelle aree interne del Paese, intraprendendo in tal modo quel percorso volto alla manutenzione del territorio e diminuendo il rischio di roghi accidentali. È importante anche la modifica della legge n. 353 del 2000, la legge quadro in materia di incendi boschivi, contenuta all'articolo 5 di questo provvedimento, che introduce la definizione di incendio di interfaccia urbano-rurale e quella all'articolo 6, che mi sta particolarmente a cuore, che interviene sul delitto di incendio boschivo, previsto all'articolo 423-*bis* del codice penale, per introdurre l'aggravante, quando i fatti siano commessi dagli addetti alla prevenzione degli incendi, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione l'interdizione dagli incarichi di prevenzione degli incendi. Rilevante è anche quella prevista dall'articolo 7, che prevede un meccanismo di premialità consentendo alle Regioni di stabilire compensi proporzionalmente incentivanti invece che in rapporto ai risultati conseguiti nella riduzione delle aree aree percorse dal fuoco, al fine di scongiurare il triste accostamento dei lavoratori precari dei Corpi forestali regionali al fenomeno dei roghi dolosi. In conclusione, era necessario aggiornare le disposizioni a contrasto degli incendi e molto è contenuto in questo decreto-legge. Per tale motivo reputo positivo il lavoro svolto dal Governo e dalle Commissioni parlamentari. Occorre, comunque, evidenziare come resti ancora vivo il problema del coordinamento tra le amministrazioni preposte e la riduzione delle tempistiche di intervento, principale causa dell'aumento delle aree distrutte dal fuoco dal 2017 a oggi. Nei fatti l'inefficace contrasto al fenomeno è principalmente dovuto alla distanza dei presidi antincendio, che incide negativamente sulla tempestività degli interventi, in aggiunta all'attuale dotazione della flotta aerea impiegata nelle operazioni di spegnimento (non si parlerà mai abbastanza del ruolo che svolgono, quasi a favore degli incendi). un maggior numero di presidi sul territorio, a garanzia di una capillarità che assicuri una risposta più rapida ed efficace. Sono certo che la sensibilità mostrata dal sottosegretario Sibilia sul tema contribuirà ad accelerare questo processo. questo processo. Ringrazio i relatori Quarto e Briziarelli per il lavoro svolto a favore di quest'Assemblea legislativa. Con questo provvedimento il fenomeno criminale che ha segnato la nostra storia recente si appresta a essere ridimensionato nel futuro, a tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e della produzione agroalimentare del nostro Paese.

che giornalmente ormai combattono gli incendi, per cercare di porre rimedio a situazioni che hanno una precisa responsabilità e che un Parlamento maturo come il nostro deve cominciare a riconoscere. Ne parlerò magari più avanti. Quello che appare evidente è l'ormai solita tendenza, tutta italica, di legiferare sull'emergenza. Tra l'altro, guarda caso, l'emergenza di questi ultimi cinque anni è legata proprio all'aumento degli incendi boschivi, che ha una precisa responsabilità: quella di essersi privati dell'unico corpo che in realtà faceva prevenzione, cioè il Corpo forestale dello Stato. Io credo che, a fronte di questo, una parte di questo emiciclo sa se oggi stiamo intervenendo anche con delle risorse, è perché allora si sbagliò la scelta.

Però mi chiedo: se non si fosse deciso con la legge Madia, durante il Governo Renzi, di privarsi del Corpo forestale dello Stato, oggi saremmo in queste condizioni?

si sbaglia di grosso, perché vorrebbe dire che un'intelligenza artificiale potrebbe sostituire i parlamentari della Repubblica. Ecco, a qualcuno piacerebbe anche, ma in realtà la democrazia è qualcosa di diverso da questo. Quindi credo che, se magari il concetto che sarebbe meglio

nazionale italiano. Non occorre aver letto il libro del fondatore del WWF Fulco Pratesi per capirlo e per saperlo. Basterebbe osservare i dati degli ultimi anni: fino a pochi anni fa la maggior parte della popolazione viveva nelle aree rurali, con tutto quello che ne consegue, cioè con la manutenzione del territorio, con il presidio, con il controllo. cento viveva nelle aree rurali e solo il 30 per cento viveva nelle città. Oggi siamo arrivati a una condizione di quasi parità. Se non si inverte il *trend*, nel giro di vent'anni avremo rovesciato le percentuali, cioè il 30 per cento vivrà nelle aree rurali, privando quindi il territorio di un grandissimo presidio, e il 70 per cento vivrà nelle aree urbane. Questo ha già un effetto,

Non servono uno studio scientifico e una visione dal satellite per capirlo, ma basterebbe interrogare le comunità locali. Prima il mio collega La Pietra l'ha detto in maniera molto chiara:

il mantenimento del territorio lo fanno i cacciatori. Fatevene una ragione! *(Applausi)*. Quel mantenimento è fatto per un equilibrio costante tra uomo e natura, tra gli stessi protagonisti della natura. natura. Criminalizzare la caccia, oppure, in maniera subdola, voler inserire un emendamento in base al quale, se c'è un incendio a Rovigo, non si caccia a Belluno mi pare quantomeno bizzarro

(qualcuno di voi più di altri) di dire: abbiamo sbagliato. Oggi dovremmo dire: ritorniamo a quel sistema che faceva prevenzione.

decise di privarsene. Ebbene, oggi, anziché votare provvedimenti *spot,* mettetevi una mano sulla coscienza e votate la proposta di legge che reintroduce il glorioso Corpo forestale dello Stato. *(Applausi)*.

sono ancora ben impresse nella mente di tutti quanti noi e in quella di moltissimi italiani, alcuni dei quali hanno assistito alla totale devastazione procurata dalle fiamme degli incendi appiccati. una situazione insostenibile che ha spinto giustamente il Governo a intervenire. È una fattispecie questa che necessitava senza dubbio un intervento legislativo straordinario e urgente per prevedere punizioni più esemplari - certo - ma soprattutto per prevenire, finanziando e sostenendo maggiormente enti locali, la Protezione civile e tutta la struttura delle componenti statali impegnate nella lotta ai roghi. prima di entrare nel dettaglio del provvedimento, vorrei esprimere la mia vicinanza e quella del Gruppo PD alle famiglie e ai parenti delle persone che in estate hanno perso la vita negli incendi, ai tanti cittadini che hanno letteralmente visto bruciare il lavoro di una vita, le proprie case e il proprio bestiame. Tutto ciò è accaduto soprattutto nel Sud Italia e, nello specifico, nelle sue aree interne, spesso già duramente segnate e colpite da mancanze di altro tipo. Quelle immagini mi hanno profondamente colpito, ma di fronte a una situazione di tale gravità la risposta delle istituzioni non può essere rappresentata dal semplice cordoglio. Serviva una risposta concreta e ritengo che il provvedimento aggiunga un importante tassello di concretezza al grande lavoro che ancora bisogna portare avanti per scongiurare episodi di natura incendiaria e dolosa purtroppo in aumento. Le direttrici su cui poggia il provvedimento si individuano nell'articolazione degli strumenti programmatori di coordinamento con le finalità di prevedere, prevenire e mitigare i rischi. Tutto ciò si rende possibile - come dicevo all'inizio del mio intervento e come vedremo a breve - rafforzando le diverse componenti operative e incrementandone le capacità di intervento. Al comma 3 dell'articolo 1 è previsto un Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento delle capacità operative finalizzato proprio alle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Una decisione che, aggiunta allo stanziamento di risorse previsto all'articolo 2 per l'acquisto di ulteriori mezzi e attrezzature, rafforza la nostra struttura e la nostra capacità di contrastare questo fenomeno. L'articolo 5 del provvedimento introduce, al comma 1, una nuova definizione di incendio di interfaccia urbano-rurale. Con questa definizione riusciamo a dare una connotazione agli incendi boschivi che interessano zone o aree nelle quali sussiste una interconnessione tra strutture che vengono definite antropiche e aree naturali. Alla luce di quanto accaduto questa estate, riuscire a individuare situazioni e aree di questo tipo ci permette di leggere meglio e prima il pericolo di eventuali incendi, ma anche di proteggere la vita delle persone potenzialmente coinvolte in questi ultimi. Da ultimo, all'articolo 6 si introducono modifiche al codice penale che prevedono da una parte aggravanti, nel caso in cui l'azione delittuosa sia commessa proprio da coloro che avrebbero invece il ruolo di prevenire gli incendi, e dall'altra attenuanti, per coloro che si impegnano a collaborare con le autorità. Esse rappresentano a mio avviso un miglioramento della disciplina preesistente. Utilizzo questi ultimi secondi del mio intervento per sottolineare l'enorme impatto ambientale che un incendio produce nel nostro ecosistema. Per questo credo siano state rassicuranti le parole pronunciate questa estate dal *premier* Draghi, che non solo ha prontamente garantito ai sindaci dei territori colpiti un programma di ristori per le persone e le imprese colpite, ma ha anche assicurato un piano straordinario di rimboschimento e messa in sicurezza degli stessi territori. Ritengo che questi impegni, insieme al provvedimento che oggi discutiamo e che ci accingiamo a convertire in legge, con un positivo contributo del Senato teso a modificare e a integrare il testo iniziale, rappresentino un significativo passo in avanti che un Governo e uno Stato civile possono fare per i propri cittadini rispetto a simili emergenze. In questa direzione dobbiamo continuare a muoverci nel futuro prossimo, affinché la vita degli italiani e la bellezza del nostro territorio non vengano inutilmente distrutte per mano di un manipolo di delinquenti. *(Applausi)*. PRESIDENTE. È iscritto a parlare

ci sono delle luci e delle ombre, a seconda del punto di vista. Mi soffermerò brevemente su una luce e su quella che sembra essere una grande ombra che caratterizza il nostro lavoro di conversione di questo decreto-legge. La luce, a mio modo di vedere, è l'aver inserito specificamente, con un emendamento a prima firma De Petris e Buccarella, a cui poi si sono aggiunte le firme dei componenti del Gruppo Misto e del MoVimento 5 Stelle, la specificazione di dotarsi, nelle prossime

per scongiurare il ripetersi di fenomeni come quelli accaduti la scorsa estate. Parlo più precisamente dell'utilizzo delle tecnologie, a cui noi spesso affidiamo tanto nella nostra vita professionale e politica, ma anche privata; tecnologie che oggi consentono, mediante l'utilizzo di radar implementati da videocamere a infrarossi e con il supporto di droni, muniti anch'essi di sensori, di poter intervenire in maniera veramente tempestiva quando ci sono gli inneschi degli incendi. È stato detto e ribadito anche qui in Aula e l'abbiamo sentito nel corso delle audizioni svolte: se è vero che le condizioni climatiche favoriscono la nascita degli incendi e la portata degli stessi agli sconvolgimenti climatici e alla siccità), molto spesso vi è anche la mano dell'uomo. Quindi noi possiamo, come abbiamo fatto giustamente, irrigidire il quadro giuridico e sanzionatorio, aumentando le pene, comprese quelle accessorie, già previste nel nostro ordinamento all'articolo 423-*bis* del codice penale. Il problema che dobbiamo però affrontare ogni volta e che adesso sembra avere portata

dolosa. Adesso è possibile fornire gli apparati dello Stato e delle Regioni di sistemi di controllo immediato e di verifica istantanea della nascita di focolai in base ai rilievi termici dei sistemi *radar,*

che si trovano nei pressi dei punti di innesco. Infatti, come cercavo di dire prima, possiamo agire giustamente su tutti i sistemi di prevenzione, tutela e rafforzamento del contrasto postumo agli incendi quando questi assumono grande scala, scala, ma se riuscissimo a impattare e punire, previa identificazione, i responsabili dell'ecocidio che ha contraddistinto l'ultima stagione estiva, faremmo un grande passo avanti nel raggiungimento dell'obiettivo. Questo è un aspetto che appare secondario nell'ambito di tutte le modifiche legislative che siamo riusciti ad apportare nel corso dei lavori in Commissione, però mi corre l'obbligo di

limitatamente alla stagione in corso, dopo eventi catastrofici per la vegetazione e la fauna dovuti ai vastissimi incendi. A mio

Ogni tentativo di mediazione è andato fallito; non possiamo che prenderne atto e riservarci la valutazione sul disegno di legge che stiamo per licenziare.

questa avventura della vita, cercheremo un riscontro per capire se le misure che stiamo adottando adesso saranno sufficienti a poter garantire quel livello di abusata - del nostro *habitat* e della nostra biodiversità forestale. Speriamo che gli obiettivi che ci siamo prefissati siano raggiunti. Qualche perplessità - a voler essere molto moderati - per quanto riguarda l'aspetto della tutela della fauna è lecito averla. Vedremo se riusciremo a vincere

detto "finalmente" perché quella che si è da poco conclusa è stata la campagna antincendi boschivi che ha registrato i dati peggiori dal 2008. In quegli anni la sensibilità generale nei riguardi dell'ambiente era sicuramente meno pronunciata di ora, e come Forza Italia, da sempre attenti alle questioni ambientali, proprio per questo motivo attendevamo questo provvedimento, che si pone l'obiettivo di arginare e ridurre i danni legati a tale fenomeno. Lo hanno già fatto i miei colleghi, ma è bene ribadire i numeri: in Italia il bosco rappresenta l'83 per cento della superficie forestale e ricopre il 29 per cento dell'intero territorio nazionale. Nonostante questo immenso patrimonio in termini di biodiversità ed ecosistemi, siamo purtroppo il primo Paese del Mediterraneo e d'Europa in cui bruciano più boschi, in particolare nelle Regioni del Sud Italia e purtroppo anche nella Regione dalla quale provengo, la Calabria, dove sono stati registrati 9.257 richieste di intervento solo quest'anno e solo in tre mesi. Il bilancio drammatico è stato di sei vittime e tanti feriti, 3.640 incendi, 395 Comuni interessati (seriamente colpite la Provincia di Reggio e molte zone del cosentino). Si tratta di dati veramente molto tristi. Durante la campagna antincendi boschivi 2021 sono andati in fumo 159.000 ettari di bosco, un quarto delle nuove foreste, praticamente le città di Milano, Roma e Napoli messe insieme: un colpo d'occhio dalla straordinaria drammaticità.

delle importanti proposte di modifica volte a migliorarne il testo? È semplice; quando va in fumo il nostro patrimonio forestale, va in fumo anche la nostra aria. A Forza Italia ciò incute preoccupazione ed anche per questo, con razionalità e dialogo, abbiamo cercato con tutti i colleghi della Commissione ambiente di apportare i giusti miglioramenti al provvedimento. Da sempre ci impegniamo per la tutela dell'ambiente, degli animali, e allo stesso modo per tutelare gli interessi degli imprenditori agricoli, seriamente minacciati e danneggiati dagli incendi; così come sono seriamente e quotidianamente minacciati e danneggiati dall'eccessiva presenza di fauna selvatica, problematica affrontata più volte anche in quest'Aula. Ancora una volta oggi abbiamo colto il grido di allarme delle organizzazioni agricole collegate al provvedimento in questione, lavorando in modo tale da scongiurarne gli effetti negativi. Il provvedimento quindi riveste importanza da diversi punti di vista: l'inasprimento delle pene per chi è responsabile di aver provocato un incendio, ma c'è anche altro; ad esempio il potenziamento dei mezzi e delle attrezzature, ai quali sono destinati 40 milioni solo per il 2021, con l'istituzione del Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa per chi combatte, molto spesso purtroppo con mezzi inidonei, gli incendi. Mi riferisco naturalmente al corpo dei Vigili del fuoco, Carabinieri forestali e Protezione civile, Forestali regionali e volontari, ai quali va tutto il nostro ringraziamento per ciò che hanno fatto quest'estate intervenendo durante gli incendi di cui tutti noi abbiamo l'immagine ancora nitida in mente. Una risposta forte quindi da parte delle istituzioni, soprattutto a chi ha cercato e cerca di delinquere provocando gli incendi. Naturalmente ancora tanto c'è da fare e tanto dobbiamo fare. Uno dei miglioramenti apportati in Commissione con un emendamento sul quale mi soffermo è quello relativo al rimboschimento. Gli ettari bruciati quest'estate, così come quelli andati in fumo negli anni precedenti, sarebbero ritornati ad essere parte del patrimonio forestale delle nostre Regioni solo dopo decenni. È un dato preoccupante. Rilevo che 159.000 ettari in meno significa meno anidride carbonica assorbita, quindi aria più inquinata per noi, per i nostri bambini e per i nostri nonni. altro dato: il carcinoma del polmone in Italia risulta la prima causa di morte oncologica in tutte le fasce di età negli uomini. Per questo abbiamo pensato di proporre l'autorizzazione ad interventi straordinari di rimboschimento compensativo delle superfici bruciate sui terreni di proprietà del demanio regionale. Ciò significa che sostanzialmente, grazie a questo emendamento che introduce un nuovo articolo, si consente alle Regioni di utilizzare terreni in disuso che dopo attenti studi antropici, anche grazie alla collaborazione di università ed enti di ricerca, andranno a sopperire gli ettari persi a causa di incendi boschivi. Così facendo si accelera il processo di ricostruzione delle superfici boscate e a guadagnarci sono soprattutto l'ambiente e le specie che lo popolano. Concludo, ringraziando ancora una volta tutti i colleghi della Commissione ambiente, la presidente, la capogruppo Gallone per il lavoro svolto, compresi i momenti un po' più concitati, i quali hanno sicuramente fatto intendere la passione con cui ognuno di noi svolge il prestigioso ruolo che ricopre.

il territorio rurale del nostro Paese, la stragrande maggioranza del territorio italiano e, in modo particolare, quel 35 per cento del territorio italiano costituito da aree boscate, un vero e proprio polmone importante per il nostro ambiente. Gli incendi costituiscono un problema pesante da affrontare seriamente, considerato che la maggior parte di questi sono di origine dolosa o colposa. È questo il punto. Nel merito:

oppure interesse a far scattare il divieto previsto dall'incendio. Di matti in questo Paese - faccio un inciso - ce ne sono! Io personalmente ho a che fare quasi tutti i giorni con quelli che mi dicono e mi scrivono che devo morire, che sono un "assassino di m...",

("bacioni", come si dice), ma è un matto! Ma a questo matto mettiamo in mano l'arma con il mirino? Ragioniamoci.

Altra domanda: in questo Paese chi fa la prevenzione contro gli incendi? Sicuramente quelli che presidiano il territorio. Abbiamo capito - la parco mania indiscriminata ce lo ha fatto capire - che il territorio abbandonato a sé stesso è maggiormente assoggettato agli incendi;

Sicuramente la prevenzione degli incendi non la fanno i cosiddetti ambientalisti salottieri che pontificano, ma non sanno cosa voglia dire fare prevenzione.

Sicuramente non sono quelli di prima - i vostri amici di qualcheduno, gli ambientalisti salottieri - quelli che vanno a fare questo lavoro.

visto il numero degli incendi, ove la fauna può fare quello che vuole indiscriminata, a cominciare dal cinghiale. La risposta al problema degli incendi è zone di protezione del cinghiale! Credo che siamo alla follia con quanto sta avvenendo nel Paese. Ringrazio anzitutto le associazioni agricole, che, quando hanno capito ciò che stava per succedere con l'emendamento sul quale abbiamo sprecato inutilmente tanto tempo in Commissione,

Ringrazio anche i colleghi delle associazioni venatorie, che hanno dato la disponibilità di parecchie centinaia di migliaia di loro iscritti, per fare sorveglianza e prevenzione. Dispiace quindi aver assistito in Commissione a proposte irrazionali e ideologiche, non solo per aumentare le zone di protezione con un automatismo di legge, ma chiaramente finalizzate, è emerso anche in qualche intervento, a raggiungere un altro obiettivo: fare una campagna politica. Vergogna! Grido alla vergogna, perché si usa il tema degli incendi per fare una campagna politica anti-attività anti-attività venatoria e anti-caccia, al punto tale che più volte è emerso il discorso del *referendum* per abrogare la caccia, cioè quel *referendum* nel quale si andrebbe a chiedere agli italiani di istituire un'intera zona di protezione per il cinghiale in tutto il Paese. Non importa, abbiamo capito che questo tema è visto in modo pregiudiziale, non in modo reale. guardate che insieme alla preoccupazione e al disagio delle associazioni agricole, pian piano sta arrivando anche quello di tanti altri cittadini italiani, che non sono interessati direttamente, ma che capiscono che su questi temi deve prevalere il buon senso, piuttosto che l'irrazionalità o i sentimenti

esautorarle da questo compito, con l'automatismo di una legge statale. Capisco il MoVimento 5 Stelle, perché loro nelle Regioni non toccano biglia. Questo lo abbiamo capito: se potessero le abrogherebbero *(Applausi)*, viste le continue brutte figure e i calci che prendono ogni volta dagli elettori, quando ci sono le elezioni regionali. Avremmo potuto affrontare anche noi un tema divisivo:

Troppo spesso la natura dell'innesco è dolosa: gesti irresponsabili che non hanno nessuna giustificazione. Per quanto si faccia sensibilizzazione verso il problema, ogni anno continuiamo a registrare incendi più o meno vasti Per quanto lo Stato faccia sforzi, dotandosi di mezzi e uomini per fronteggiare le fiamme e spegnere gli incendi, il danno che contiamo ogni volta rimane immane. Per ristabilire le condizioni ecosistemiche di un bosco distrutto occorrono venti anni di cure e significative risorse per ridurre il rischio di una nuova distruzione. Il problema è destinato a crescere, visti i cambiamenti climatici che stiamo vivendo e che portano stagioni estive ormai sempre più spesso siccitose e caldissime. Questa estate torrida ha confermato il *trend* e ha fatto registrare una quantità di incendi mai vista prima: migliaia, di cui circa 400 di grandi proporzioni, cioè di oltre 30 ettari ciascuno. cento della superficie italiana è coperta da boschi, una ricchezza che richiede tanta attenzione, più volte e da tante parti invocata, dal momento che gli ultimi anni hanno testimoniato una costante e inesorabile crescita. Nel rapporto sulla prevenzione e gestione forestale dell'Unione nazionale Comuni, Comunità ed Enti montani, nell'aggiornamento ad agosto 2021, troviamo che già il 2017 fu un anno terribile per gli incendi, con più di 162.000 ettari coinvolti. Siamo in ritardo. La gravità dei danni che gli incendi provocano deve necessariamente far mettere in campo tutte le soluzioni necessarie e utili a ridurre questi disastri. Purtroppo questi accadimenti sono anche troppo spesso incredibilmente alimentati dall'uso irrispettoso dei nostri boschi, da interessi criminali e, non ultimi, dall'accensione dei residui agricoli o, addirittura in aree protette, dall'utilizzo di *barbecue* o dalla disinvoltura di incauti fumatori; pratiche sconsiderate e una maleducazione piuttosto diffusa, che vanno debellate attraverso pene severe e campagne di informazione sulla dannosità per l'ambiente di qualunque combustione e sull'importanza dei boschi e dell'ecosistema che rappresentano. indispensabile e necessario per un contrasto più efficace, innanzitutto in termini di prevenzione e ovviamente di intervento, ma anche per una rapida individuazione dei responsabili di tali disastri termini di inasprimento delle sanzioni. L'incremento di risorse per mezzi e uomini, come per la ricerca di nuove soluzioni tecnologiche, è ovviamente indispensabile, ma con la consapevolezza che la prevenzione è sempre meglio della cura. È su questo fronte che la collaborazione di ogni ente, pubblico e privato, delle imprese agricole e forestali, di tutti i cittadini può essere determinante per la salvaguardia di un patrimonio, quello che la bellezza del paesaggio boschivo rappresenta. A tale proposito, nel campo degli interventi volti alla valorizzazione del paesaggio, è fondamentale il miglioramento della viabilità forestale. Bisogna prevedere un piano di rivalutazione di tutti quei percorsi antichi di mobilità lenta, fatta di strade rurali, strade bianche, tratturi, percorsi pedonali e mulattiere, che rappresentano un valore storico di rilievo e un modo per attivare nuove forme di economia locale, con cui sperimentare progetti che intersecano agricoltura, ecologia, turismo e servizi alle comunità. Ho appreso con piacere che un mio ordine del giorno è stato accolto: un impegno al Governo per interventi mirati per una strategia forestale volta alla rivalutazione di vasti areali boschivi, spesso lasciati all'abbandono, mediante la riscoperta e la valorizzazione della ruralità, del cicloturismo, del *trekking*, del turismo equestre, dei percorsi che nutrono il corpo e lo spirito. Ringrazio la presidente Moronese della Commissione territorio, ambiente, beni ambientali e i relatori Quarto e Briziarelli per il grande lavoro di sintesi tra tutte le proposte giunte, condotto con passione e diligenza. Credo che usciremo da questi eventi così deleteri per la natura e il paesaggio soltanto con azioni proattive, combinate a una capillare informazione, promozione e sviluppo, volte al rispetto per la nostra madre Terra, con i suoi boschi e la sua biodiversità, che è vita per tutti e che, quindi, non può che rappresentare un bene prezioso per i territori che possono fregiarsi della sua ricchezza. Una bellissima cornice alle nostre passeggiate, ai nostri borghi, alle nostre città,

una nuova finestra"). La Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che la seduta di domani avrà inizio con il seguito della discussione del disegno di legge in materia di contrasto della discriminazione o violenza per sesso, genere o disabilità, approvato dalla Camera dei deputati. Successivamente si proseguirà nella discussione del decreto-legge sugli incendi boschivi.